Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico:* «Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori» Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 4 febbraio. Nella seduta pomeridiana di oggi proseguirà la discussione del disegno di legge concernente le cure palliative e le terapie del dolore. Il disegno di legge comunitaria 2009 sarà posto all'ordine del giorno a partire dalla giornata di domani. Il calendario della settimana corrente è inoltre integrato con l'esame di una relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernente l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche. In apertura della seduta pomeridiana di domani, la Presidenza commemorerà la Giornata della memoria. I rappresentanti dei Gruppi potranno successivamente intervenire per 5 minuti ciascuno. La prossima settimana, con inizio dalla seduta pomeridiana di martedì 2 febbraio, sarà dedicata alla discussione dei decreti-legge in scadenza in materia di protezione civile e proroga termini legislativi. Per la ripartizione dei tempi tra i Gruppi si è seguito un criterio non strettamente proporzionale che ha tenuto conto delle richieste dei Gruppi di opposizione. Nella seduta pomeridiana di giovedì 4 febbraio saranno svolte interrogazioni a risposta immediata con trasmissione diretta televisiva per la durata di un'ora. Infine, la Presidenza ha illustrato ai Capigruppo un progetto tendente a introdurre la firma elettronica per la presentazione degli atti parlamentari, con graduale superamento della trasmissione in forma cartacea. La prima fase sperimentale, alla quale saranno chiamati a partecipare alcuni senatori indicati dai rispettivi Gruppi, riguarderà gli atti di sindacato ispettivo.

dei tecnici della Commissione, del Ministero della salute e del Dipartimento per le tossicodipendenze. Come Come ha detto la collega Baio, la società con questa legge si fa carico di chi è in una condizione di dolore. In particolare, abbiamo cercato di definire quegli aspetti che dovevano essere caratterizzati dalla precedente legge.

famoso e famigerato ricettario in triplice copia, spesso non rintracciabile, su cui il medico di base esclusivamente poteva riportare - in maniera anche complessa tutte le prescrizioni di sostanze stupefacenti, con una serie di procedure a carico

dell'organizzazione - finalmente - delle reti delle strutture palliative e delle reti della terapia del dolore: due reti distinte, ma coordinate con unità dipartimentali a livello nazionale, regionale

in ultima analisi, una rete di questo tipo non solo rende un grande servigio al malato e alla famiglia nel momento più difficile della vita,

dei farmaci per il dolore, che prima di questo intervento vedeva l'Italia nei Paesi dell'OCSE, al penultimo posto, davanti alla Grecia; Grecia; era evidentemente una situazione da sanare. Contempla inoltre la presenza delle reti delle cure palliative e delle terapie del dolore,

come un dono importante che il Parlamento e il Governo fanno al nostro Paese. È quindi con soddisfazione che ci approntiamo al varo di questo disegno di legge.

concernenti diritti sociali in materia sanitaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti,

esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "Ministero della salute," inserire le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'articolo 2, comma 1, e sull'articolo 10, comma 1, lettera *d)*. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 5.21, 5.24. 5.204, 10.0.214, 5.201, 5.202, 5.203, 10.203 e 12.200 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

al quale viene poi imposto l'obbligo di distruggere questa *cannabis*. Siccome in Italia non esistono delle case farmaceutiche che hanno fatto richiesta di produrre medicinali a base di *cannabis*, con questo ordine del giorno facciamo una proposta operativa e offriamo un suggerimento e una soluzione a quei malati che, attualmente, possono utilizzare farmaci a base di *cannabis* e sono, però, costretti a una trafila burocratica complicatissima, cioè all'importazione dall'estero.

tra le sue varie missioni, porta avanti anche le attività congiunte di ricerca e di formazione per la produzione di medicinali orfani, è è autorizzato alla produzione di farmaci e può acquistare, impiegare e distribuire sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni.

è nata una polemica in provincia di Trieste sul fatto che, per la mancanza di personale, le donne non hanno potuto accedere accedere al parto indolore. Penso che si debba garantire a tutte le donne che ne fanno richiesta la possibilità di partorire senza dolore, di poter vivere il momento di dare alla luce un bimbo in maniera tranquilla, serena e sicura. L'ordine del giorno impegna il Governo a far sì che le Regioni

clinica, tutti cattolici, tutti di destra e tutti contrari all'utilizzo della *cannabis* per altri motivi e altri scopi. Su questo tema dovremmo entrare nella sofferenza, al di là - ripeto - degli studi scientifici.

all'ordine del giorno G102, che mi sembra assolutamente di buon senso. Paghiamo un istituto che potrebbe dare benefici ai nostri malati, e lo paghiamo perché lo paga il Ministero dell'agricoltura; contemporaneamente, però, dobbiamo buttare tre quarti del lavoro che fa

Mi rivolgo alle schiene di molti miei colleghi di maggioranza, i quali, facendo in questo momento da testuggine al Ministro, gli consentono di essere distratto più di quanto dovrebbe.

che deve aver letto poco e capito evidentemente anche meno. Come lor signori notano, anche i miei tentativi di insolentire il Ministro della salute non sortiscono alcun effetto. Il che mi conforta perché, dal momento che stiamo parlando di anestetici, evidentemente è anestetizzato a tutto.

riflettano se votare a favore di questo banale ordine del giorno, il quale impegna il Governo semplicemente a valutare l'opportunità e la fattibilità di una produzione in Italia di farmaci a base di *cannabis*.

per rivolgere un appello al relatore e al Governo a svolgere un'ulteriore riflessione. Aggiungo un elemento che è stato menzionato, ma non sottolineato a sufficienza:

G102 non dice di liberalizzare la produzione di *cannabis* in Italia, ma di autorizzare due istituti pubblici,

prima di questo chiederei al relatore e al Ministro del mio Governo di riflettere qualche secondo in più prima di esprimere un parere negativo su di

In varie occasioni, anche in Commissione, si è parlato, secondo me in maniera decisamente eccessiva, di un aspetto che, nell'ambito di una legge ampia e vasta, va ricondotto al contesto originario.

inviterei a leggere attentamente la normativa vigente, cioè il Testo unico n. 309 del 1990, riguardante la regolamentazione delle terapie con sostanze stupefacenti. All'articolo 26

salvo che per scopi scientifici, didattici e sperimentali. Quindi, ci troviamo di fronte ad una normativa in essere che vieta assolutamente la coltivazione per motivi diversi da quelli esplicitati, compresi i motivi terapeutici. Un altro elemento che abbiamo tenuto in considerazione in maniera molto approfondita in Commissione è proprio quello dell'utilizzo terapeutico delle sostanze riconducibili alla *cannabis*, cioè i derivati.

sono due: il delta-8-tetraidrocannabinolo e il delta-9-tetraidrocannabinolo. Per quanto concerne il delta-8, è stato ribadito, condiviso, analizzato e studiato in Commissione quanto anche i tecnici del Dipartimento

su di esso già il ministro Turco era intervenuto (nessuno si sente qui di contraddirlo) spostandolo di tabella e inserendolo nell'apposita tabella II, sezione B, concedendone quindi totalmente l'utilizzo, come è scientificamente corretto (non entro ulteriormente in questa disamina). Detto ciò, sarebbe una situazione veramente originale, esclusivamente per questo tipo di prodotti, tirarli fuori dal contesto della normale situazione di produzione farmacologica (in cui tutte le sostanze sono prodotte normalmente dall'industria farmacologica e di solito senza grande

sulla terapia del dolore e ricordo tutti coloro che hanno lavorato nei vari schieramenti, così come i tanti e tanti emendamenti

presa in carico da parte dello Stato e del Servizio sanitario nazionale di questa grave situazione. Per questo motivo, con molta serietà e convinzione (vedrete che il successivo testo lo confermerà), ribadisco il mio parere

D'altro canto, non esistono ancora oggi in prontuario terapeutico dei farmaci normalmente commercializzati con il delta-9-tetraidrocannabinolo, mentre sono stati inseriti all'interno della tabella ministeriale

per aver preso in considerazione la possibilità che l'Assemblea si esprima liberamente su tale ordine del giorno; ringrazio altresì il senatore Saia e in particolare il presidente Baldassarri, che ha dato l'interpretazione autentica di ciò che tale ordine del giorno chiede.

Non si tratta di andare contro la legge del 1990, tanto che il relatore, poco fa, ha ricordato che all'interno di tale legge è consentita la produzione per motivi medico-scientifici e di ricerca. un impegno del Governo a valutare l'opportunità e la fattibilità di una produzione, già autorizzata in Italia, di farmaci a base di *cannabis*, grazie a strutture pubbliche

proprio perché siamo coscienti del fatto che ogniqualvolta si parla di determinate sostanze o piante (all'interno della Convenzione del 1961 delle Nazioni Unite) si ha a che fare anche con le leggi che poi hanno inglobato a livello nazionale quelle norme, c'è il problema

la possibilità di valutare l'opportunità e la fattibilità di una produzione di principi che da studi internazionali sono inclusi nella varie terapie del dolore per quanto riguarda il dolore neuropatico, tumorale, da emicrania, da sindrome di Tourette, glioblastomi e da artrite reumatoide. Ripeto, noi non vogliamo che da domani si produca questo in Italia. Chiediamo che si possa prendere in considerazione il fatto che i malati italiani non siano

La nostra preoccupazione è evidente: non vorremmo che passasse una posizione a favore di una legalizzazione

superando anche il problema creato da un mutamento di opinione del Governo nella indicazione del suo atteggiamento nei confronti dell'Aula. *(Applausi

Il dibattito svolto la settimana scorsa sulle questioni generali affrontate da questo disegno di legge non ha preso in considerazione (forse anche perché figlio di tempi molto ristretti per la presentazione dei documenti)

seppure in alcune parti ancora tutta da interpretare, della legge che ha a che fare con le cure del dolore in virtù dell'architettura internazionale che regolamenta in maniera molto stretta offerta e domanda legale (quindi non offerta e domanda reale). Siccome

italiana non consentirà di approvvigionarci delle quantità necessarie derivanti da questo grande aumento della domanda reale che automaticamente l'Italia certificherà alle Nazioni Unite come domanda legale.

questo caso non starò a chiedere una sospensione per una nuova discussione. Bisognerebbe però capire se, in effetti, il Governo è al corrente del problema che si andrà a presentare il giorno dopo in cui questa legge entrerà in vigore: in vigore: ci dovremo presentare alla Commissione narcotici di Vienna chiedendo anche la centuplicazione delle quote di morfina, per esempio, da comprare in virtù di questa nuova legge. Questi ci diranno che non è possibile perché la nostra domanda legale

una serie di accorgimenti, mentre il diritto è qualcosa che si può poi utilizzare meglio.

1.3. Ancora una volta capisco che si voglia far uscire senza modifiche questo provvedimento dal Senato, però l'emendamento 1.3 chiede di aggiungere al comma 2, dopo le parole «terapia del dolore»,

va nella direzione di quello che un legislatore dovrebbe fare, cioè richiamare la possibilità che i diritti vengano goduti da persone che in questo caso sono anche malate. Infatti, al comma 2, si chiede di sostituire le parole «bisogno di salute» con

2.2 torna a ribadire un concetto che avevamo cercato di inserire nell'articolo 1, cioè che accanto alle terapie del dolore apparissero anche le di altre cause di sofferenza, sempre per cercare di approvare una legge il più fruibile possibile, fruibile dal maggior numero di persone. Ed in questo caso si sta parlando di pazienti.

la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita». Entriamo così tanto nello specifico che temo che una persona malata

è la persona affetta da una patologia. Non andiamo oltre, non specifichiamo altro, perché poi davvero c'è il rischio che, una volta che questa legge venga pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, qualcuno ne resti fuori

È stata fatta una lunga enumerazione di cosa si intenda per dolore, ma molto probabilmente non si è esaustivamente trattato, malgrado i lavori anche alla Camera, cosa possa portare dolore o sofferenza. Questo è il minimo cambiamento che vorremmo si introducesse. Per questa ragione chiedo che tale emendamento

un catalogo di possibilità contestuali. Capisco che si sia fatto un grande lavoro ed uno sforzo anche "creativo" nel tentativo di descrivere di cosa si tratta, ma secondo noi meno si approfondisce e più si va incontro

era cogente nei confronti delle Regioni che disapplicavano la legge. Vi leggo la norma che abbiamo cancellato: «Nel caso in cui una Regione ritardi o ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, fissa nei confronti della Regione inadempiente un termine ultimo per la realizzazione dei dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, in caso di perduranza dell'inadempimento si applica l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi di cui alla presente legge». In altre parole,

(alcune sono più rispettose di come vengono utilizzati i fondi, altre un po' meno), credo che questo comma sia davvero importante. Questo è il senso dell'emendamento 3.200.

in virtù del fatto che si introduce un nuovo meccanismo che potrebbe creare ulteriori necessità di fabbisogno economico, non si voglia prevedere

non si fa altro che confermare una decisione importantissima in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni regionali.

canto, con l'emendamento del relatore, introduciamo ancora una volta (come se fosse necessario farlo) il concetto che il Ministero della salute deve concertare tutto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

il sistema sanitario nazionale? Noi abbiamo già condotto una battaglia, quando è stato istituito il Ministero della sanità, per non creare questa sudditanza rispetto al Ministero dell'economia. Ribadiamo questo principio e ribadiamo con forza che vogliamo che

si impone alle Regioni che non assolvano ai loro obblighi almeno di non usare le risorse a loro totale discrezione, senza fornire

«all'effettiva presa in carico del malato da parte del Servizio sanitario nazionale ed alla continuità dell'assistenza». Le parole, in una legge, devono essere chiare e devono far scattare diritti e doveri.

razionalizza e modifica profondamente i contenuti di questa legge, che in tutti i suoi passaggi prevede esclusivamente la formazione di due reti, una della terapia del dolore e una

per sottoporsi alla terapia del dolore. Credo che una razionalizzazione di queste due reti in un'unica organizzazione perlomeno dipartimentale, o quanto meno stabilire che all'interno delle singole strutture sanitarie queste due branche lavorano congiuntamente

non solo rispetto agli altri Paesi europei ma anche in termini di disomogeneità da regione a regione. È stato messo in risalto anche da dati del Ministero della salute che, a fronte di una rete di *hospice* di circa 120-140 strutture,

Nel momento in cui si procederà ad un monitoraggio della situazione delle strutture deputate alla medicina palliativa e alla terapia del dolore e si procederà ad una rilevazione

quella della medicina palliativa e quella della terapia del dolore, ma anche alla necessaria uniformità territoriale nella redistribuzione di questi servizi essenziali, in maniera da porre

5.29 ha costo zero perché, fermo restando l'importo complessivo delle risorse messe a disposizione per l'integrazione delle due reti di medicina palliativa e di terapia del dolore,

come indici il numero degli abitanti delle singole Regioni e anche il livello di mortalità in relazione alle malattie neoplastiche o croniche degenerative. A questi criteri aggiungiamo anche un'altra specificità. In sostanza, proprio per colmare quel *gap* tra alcune Regioni a livello zero di assistenza ai malati terminali rispetto ad altre che

del bisogno di dare una uniformità di assistenza agli italiani, tra i vari criteri poniamo anche l'indice della presenza, maggiore o minore,

Signora Presidente, abbiamo presentato una serie di emendamenti perché siamo convinti che le cure palliative e le disposizioni per poterle realizzare necessitino anche di un'organizzazione territoriale adeguata. Siamo quindi convinti che un disegno di legge debba dare qualche linea nella direzione di garantire le migliori competenze e la migliore organizzazione territoriale per potersi realizzare; altrimenti rischia di essere in qualche modo solo una bandiera. in sintonia anche con quanto prima proposto dal senatore Rizzi, da una parte proponiamo una articolazione territoriale di unità semplici e complesse con collegamenti dipartimentali, per poter garantire l'organizzazione territoriale di queste unità per le cure palliative per la terapia del dolore; dall'altra parte, introduciamo un concetto di competenza del personale che andrà poi a far funzionare dette unità.

perplessità o comunque un motivo ostativo da parte della Commissione bilancio, chiederei in qualche modo la possibilità di accantonarli per una eventuale riformulazione compatibile il superamento dei problemi posti dalla stessa Commissione bilancio. Ciò anche perché è chiaro che la proposta si svolgerebbe nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili per le spese del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.27, anche noi nutriamo la preoccupazione che i servizi non siano uniformemente erogati sul territorio, non solo in termini di qualità e quantità, ma anche di costo. introduciamo l'idea di un tariffario nazionale che regoli le prestazioni su tutto il territorio, per omogeneizzare al massimo i costi e, quindi, la presenza delle prestazioni in tutte le Regioni, nelle quali oggi si registra invece una grande disomogeneità.

la possibilità di partorire con minore dolore e con una più attiva partecipazione da parte della donna ci pare estremamente coerente con uno dei principi del provvedimento in esame; oggi purtroppo questo non avviene.

non credo che questo cambi le sorti del mondo. Il Presidente della Commissione sanità, che è anche un ginecologo, scuote ora la testa per dire che sicuramente incide dal punto di vista economico. Ci mancherebbe! Non è per opera dell'acqua santa che noi possiamo intervenire sul processo del travaglio di una donna. Io credo che questa sia l'occasione. Signor Ministro perché lo perché lo rifiutiamo? Io vi chiedo di ripensare un attimo: si tratta di scegliere ed è una scelta di civiltà che all'interno dei Paesi europei

Presidente, potrebbe il Ministro spiegarci? Mi rivolgo al Ministro della salute in Italia e mi domando se, in un provvedimento di questo genere, che prevede tutta una serie di cose per alleviare il dolore,

davvero importante. L'altro aspetto del problema è quello di creare un gruppo di professionisti che possano assistere tali pazienti; quindi occorre una formazione adeguata

a un bisogno fortemente sentito dai malati, (un'efficace terapia di contrasto del dolore, in particolare nelle fasi descritte nella legge) e da tutto il mondo scientifico, visto che è una pratica prevista in tutto il mondo. Siamo però convinti, colleghi, che non basta approvare una legge perché le cose si realizzino. Ripeto l'esempio che faceva poco fa il presidente Ignazio Marino: c'è la legge sugli *hospice*, ma poi ci sono Regioni in cui gli *hospice* esistono e Regioni in cui non ce n'è neanche uno. Ciò che viene stabilito con questo emendamento - il testo licenziato dalla Camera prevedeva un osservatorio, ma lo strumento in questo momento non è importante: importante è la funzione che il Governo sia in grado di ottenere tutte le informazioni dalla Regione (e naturalmente di scambiare informazioni con le Regioni) per poter avere un monitoraggio costante dell'applicazione della legge,

e al Ministro: questa non è una legge che serve soltanto per dire che ne abbiamo approvata una, ma è una legge che dovrà essere trasformata in pratica clinica e in attenzione ai pazienti e richiede un impegno del Governo a monitorare i risultati e a riferire in merito

utilizzare non soltanto il ricettario speciale, quindi non soltanto la cosiddetta ricetta rossa del Servizio sanitario nazionale, ma anche la ricetta

Se parliamo di farmaci, se parliamo di una legge che interviene a favore dei pazienti e di persone che hanno bisogno di cure, credo che il Dipartimento per le politiche antidroga possa essere tranquillamente tenuto fuori.

A me non interessa entrare nello specifico della cultura antidroga, perché credo che le esperienze politiche di ognuno di noi siano storicamente così limpide, chiare e adamantine e adamantine da non poter essere messe in discussione. Credo di far parte di una generazione politica che ha fatto su questi temi delle battaglie, spesso solitarie, nella propria esistenza, con molta chiarezza.

A me interessa anche sottolineare un'altra cosa. L'ho già detto prima. Vengo da una famiglia di medici e non voglio mettermi a far la gara sulle qualità di chi è contro e di chi a favore su questi argomenti. Non mi interessa neppure, perché non sono competente su questa materia, ragionare sui testi e sugli studi scientifici sulla materia, perché su tanti altri argomenti, su tanti altri farmaci e su tante altre questioni relative relative alle terapie, non solo del dolore, ci sono disquisizioni che durano anni e anni, dove si contrappongono teorie e tesi diverse. Non mi interessa questo (e mi riferisco in particolare ad una

riescono ad avere una qualità della vita sufficiente per poter ancora vivere, per scacciare la voglia di farla finita (lo dico con chiarezza); quando ci sono medici che su questo tema hanno posizioni favorevoli (non m'interessa se poi ci sono altre tonnellate di studi scientifici che mi dicono il contrario). Non mi interessa entrare all'interno delle dinamiche farmaceutiche se in Italia non c'è interesse a produrre questa tipologia di prodotti perché vi è una bassa richiesta; non mi interessa discutere se noi qui dobbiamo dare inizio alla coltivazione: nessuno vuole questo (almeno, sicuramente non lo voglio io). Ma ci sono Paesi in cui è vietato tanto quanto in questo Paese l'utilizzo di sostanze stupefacenti a uso ludico - l'Austria, la Gran Bretagna, il Canada, gli Stati Uniti e la Germania - dove questi

e a superare i crampi alle gambe, alla schiena, la difficoltà di respirare di notte, con l'intervento di pronto soccorso con una regolarità purtroppo unica, riesce ad avere una qualità della vita diversa con un farmaco che si chiama Satirex, una

anche nella tabella II: quindi è un farmaco prescrivibile. Non capisco perché può esserci la morfina e non può esserci questo derivato dalla *cannabis*. Ciò non significa aprire le frontiere all'utilizzo delle droghe in questo Paese. Lo voglio rispecificare mille volte. Non si può ragionare con l'accetta su questi argomenti. Credo mi comprenda solo chi ha vissuto esperienze che ti portano a stare in mezzo ai malati che ti guardano con gli occhi disperati dicendo di fare qualcosa

a tanto al chilo gli studi scientifici che si contrappongono a questo o quell'altro. Ciò non significa assolutamente aprire all'utilizzo di sostanze stupefacenti nel Paese: si tratta semplicemente di

definibile politicamente e sul piano tecnico come apertura all'utilizzo delle droghe.

chiave importante di questo disegno di legge. Non possiamo parlare di terapia del dolore e di unità di cure palliative organizzate sul territorio, né possiamo parlare di continuità territoriale, sanitaria e socio-assistenziale,

nell'emendamento 10.202, introduco il concetto che il ricettario del Servizio sanitario nazionale, che rappresenta un passo in avanti nella semplificazione dell'uso di questi farmaci, possa essere distribuito non solo ai medici di medicina generale, di pediatria, di base o agli specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ma a tutti i medici operanti, a qualsiasi titolo, nel settore delle cure palliative e della terapia antalgica. Sappiamo che ci sono tanti medici che lavorano in ONLUS e in associazioni che curano i pazienti a domicilio e, secondo me, sarebbe giusto semplificare la vita sia a questi operatori della sanità, sia alle famiglie che ospitano a domicilio pazienti in stato terminale,

nell'ambito della legislazione di settore, non affrontando soltanto aspetti di tipo tecnico, ma trattando un problema di natura culturale. Non vi

del principio di cautela, secondo il quale potenzialmente il paziente può essere un tossicodipendente e tutti gli operatori della sanità possono essere dei potenziali narcotrafficanti. ma è per indicare la prevalenza di un sistema di vigilanza, di controllo e di contrasto incalzante attraverso norme stringenti, che hanno determinato dinanzi alla strada del paziente, del medico e del farmacista, un labirinto del quale poi ci si perde. Questa legge mette la parola fine a questa situazione ed inverte: rigore, rispetto delle norme, monitoraggio, elementi di tutela e di garanzia per i corretti livelli di accesso alla terapia,

Credo che alcuni aspetti tecnici contenuti soprattutto in questo articolo 10 non abbiano consentito anche ai colleghi

De Lillo, che l'attività emendativa del Senato ha concesso di evitare alcuni problemi al testo licenziato dalla Camera. Voglio dirlo soprattutto ai colleghi Bosone e Cosentino:

i criteri per la formazione della tabella delle sostanze stupefacenti; nulla ha a che fare quella parte che volete emendare, facendo un salto indietro e recuperando il testo della Camera, sul versante della facilitazione, della semplificazione all'accesso, aspetti questi che sono normati dagli articoli 38, 43 e 45, che riguardano appunto le modalità di prescrizione e di dispensazione. Questo vorrei che fosse chiaro, perché vale la pena che si riconfermi su questa legge un convinto parere positivo, che trova riscontro non soltanto attraverso gli emendamenti già approvati in Commissione, ma anche attraverso gli emendamenti che con alcuni colleghi ho sottoscritto e che creano condizioni di controllo necessario sull'attività di distruzione degli stupefacenti, allorché non più utilizzabili,

a beneficio dei medici che operano in questo settore presso strutture sanitarie private e pubbliche accreditate con il Servizio sanitario nazionale; gli obblighi della conservazione della documentazione e di omogeneizzazione (si riporta tutto a due anni come obbligo di conservazione); la depenalizzazione delle violazioni formali formali (le attuali sono palesemente collidenti con il principio della congruità della sanzione). Insomma, signor che gli emendamenti - sui quali, ove dovesse essere necessario, nello specifico sono disponibile eventualmente a ritornare per portare un ulteriore contributo servono a concludere l'*iter* procedimentale di questo disegno di legge (che sarà salutato, come già sta avvenendo in queste ore, dalla comunità nazionale, nazionale, dai pazienti e dalla comunità scientifica con ogni forma di apprezzamento), così come noi abbiamo tentato di fare nel lavoro che sin qui abbiamo svolto. *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, alcuni dati del nostro Paese. Ogni anno ci sono 250.000 persone che muoiono per malattie considerate inguaribili. i dati ci dicono che per il 58 per cento dei malati che provano dolore non vi è nessun controllo del dolore dei casi, quindi quasi sette su dieci, vengono prescritti farmaci che sono considerati assolutamente inadeguati dall'Organizzazione mondiale della sanità. In pratica, nel nostro Paese, tra i pazienti che soffrono per dolori a volte atroci, solo il 9 per cento riceve oppioidi deboli e solo poco più dello

che ogni medico, abilitato a seguire dei malati perché abilitato alla professione, possa prescrivere i farmaci per il dolore e lo possa fare come avviene, con meccanismi stringenti, in Paesi che hanno norme e regole severe. Questa, che certamente non potete vedere perché siete distanti, è una fotocopia del mio ricettario negli Stati Uniti. È un ricettario bianco, che viene consegnato al farmacista, il quale prende il nome del medico, il nome del paziente e lo trasmette alla DEA, l'agenzia che controlla gli oppioidi negli Stati Uniti. Nell'emendamento in questione, io propongo una norma ancora più stringente: che il farmacista riceva la ricetta, che dia il farmaco in modo che il paziente ne possa trarre beneficio e che, ogni trenta giorni, trasmetta all'Ordine dei medici e all'ASL quella ricetta.

che questo emendamento non venisse accettato: il professor Umberto Veronesi non potrebbe prescrivere su un ricettario 10 milligrammi di morfina per un suo paziente terminale. Insomma, è ovvio che non è questo il modo di procedere per una legge con la quale vogliamo portare aiuto

possono distruggere gli oppioidi che rimangono nei loro magazzini affidandosi praticamente ad aziende private e facendo un verbale senza nessun controllo. In pratica, quindi, approvando la legge così com'è, noi possiamo avere, da un lato, lo smaltimento di decine di fiale di di morfina senza alcun controllo, ma il professor Veronesi non può prescrivere dieci milligrammi di morfina a un malato oncologico che muore di dolore. Davvero dobbiamo metterci la mano sulla coscienza nel votare questo emendamento. Chiedo molta attenzione soprattutto a quei senatori, come il senatore Saia e il senatore Saro e a tutti i medici della maggioranza, a partire dal presidente della Commissione igiene e sanità, senatore Tomassini, e al Ministro della salute, che è medico. medico. Semplicemente, noi dobbiamo approvare una legge che consenta a tutti i medici di prescrivere i farmaci per il dolore con controlli rigorosi e severi.

Certamente, però, lo abbiamo affrontato anche nel momento in cui abbiamo ricevuto questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, con l'intento di migliorare addirittura la possibilità di fruizione, anche degli oppioidi, da parte di tutti gli ammalati e di tutti coloro che sono colpiti colpiti dal dolore. Certo, è molto pietoso, molto importante, delicato e vicino il dolore, così come lo ha raccontato il collega Saia,

Ma quanti passi avanti con questa legge si compiono nell'andare incontro al malato! La semplificazione delle norme, già prevista dalla Camera, non viene per nulla diminuita dalle modifiche che attentamente la Commissione igiene

Signor Presidente, non è una questione ideologica quella che stiamo toccando in questo momento. Vorrei quindi pacatamente riflettere insieme all'Aula, indipendentemente dalle distinzioni di schieramento. Il tema è il seguente: soltanto i medici abilitati all'uso del ricettario speciale, del ricettario rosso delle ASL, o tutti i medici possono prescrivere, per esempio, per esempio, la morfina ai propri pazienti che hanno il problema di avere una capacità di risposta ad un dolore spesso drammatico? Vogliamo o no consentire ai medici, che sono tutti abilitati all'esercizio della professione, il diritto di prescriverla? Se diciamo di sì e riconosciamo la loro professionalità e il loro valore, abbiamo bisogno di norme rigorose per evitare abusi. E infatti il farmacista deve inviare tutti i mesi queste ricette all'ordine dei farmacisti e alla ASL, poi l'ordine dei farmacisti ne reinvia un sunto al Ministero nei quindici giorni successivi. È un controllo da cui non si scappa, perché la ricetta è firmata

Si può obiettare che non siamo sicuri che non vi saranno abusi, ma il sistema di regole è molto efficace, molto più efficace, ad esempio di quella norma che veniva invece già ricordata dal collega Marino, in cui si prevede la distruzione di decine o centinaia di fiale di morfina sulla base della pura redazione di un verbale. Per colmo

Allora, se si lasciano le cose come stanno e non si riesce a regolare bene neppure la distruzione, perché non si pensa invece che sia molto più efficace il controllo nella prescrizione fatta inviando tutti i mesi, sia alla ASL, sia all'Ordine dei farmacisti, le ricette che sono La verità è una sola, colleghi: in linea di principio, non si vuole riconoscere ai medici un diritto che si sono conquistati con la loro professionalità, cosa che non fanno per se stessi, ma per i loro assistiti. Non c'è una ragione pratica per dire di no,

avremmo dovuto trovare un clima e un livello di pacificazione in nome della gente che, a causa

Avendo ricevuto un parere negativo, l'esito mi pare scontato. Spero, però, grazie anche al dibattito scaturito dalla riproposizione di questi emendamenti, che alcune delle zone grigie - molto scure per quanto ci riguarda e magari più chiare per la maggioranza - che questa legge porta con sé verranno affrontate a seguito delle dichiarazioni rese dagli esponenti del PdL in Aula. Auspico quindi che si faccia grande pubblicità a questo dibattito che, grazie a detti emendamenti, è venuto fuori, perché in qualche modo si andranno ad aiutare i medici

A loro va il saluto dell'Assemblea.

credo sia utile che questo dibattito riporti a più voci l'importanza di separare e scollegare l'uso ludico che si può fare di una sostanza rispetto all'uso medico e terapeutico della stessa. della stessa. Chi è medico sa bene che di una stessa sostanza come - per esempio - il papavero da oppio si può fare un uso con l'eroina e un altro con la morfina. Probabilmente la parola *cannabis* tende a sovrapporre due usi così diversi come quello ludico e ricreativo e quello medico e terapeutico.

In questo momento, però, vorrei anche ricordare che cosa succede oltre oceano e che cosa è successo dopo che alla Casa Bianca vi è stato il cambio dalla Presidenza Bush alla Presidenza di Barack Obama.

C'è però uno Stato federale che, a differenza dell'Italia, non prevede l'obbligatorietà dell'azione penale e prevede che la politica federale, attraverso l'FBI, segua indirizzi politici.

Con la Presidenza di Barack Obama è cambiato semplicemente l'indirizzo politico dato al Ministro della giustizia. Stati americani - l'Alaska, la California, il Colorado, le Hawaii, il Maryland, il Michigan, il Montana, l'Oregon, il Rhode Island, il Vermont e Washington - che durante gli otto anni della Presidenza Bush avevano visto violata la possibilità che le loro leggi statali

il principio attivo della *cannabis* terapeutica è stato inserito nella Tabella II attraverso un decreto del ministro Turco nel 2007, anche

in virtù del fatto che l'emendamento successivo, il 10.203, è - a parer mio - pressoché identico, mentre a parere della Commissione bilancio evidentemente no, dato che è stato giudicato negativamente dalla stessa Commissione. Comunque, l'importante è salvare la sostanza

Presidente, mi perdonerà se in altre occasioni sono intervenuto diciamo in modo irrituale, però credo che ci siano dei momenti nei quali la polemica politica anima il dibattito ed altri momenti nei quali diventa strumentalizzazione assolutamente oziosa, un esercizio che ci allontana dal conseguimento dei risultati. Poi ci si chiede perché la piazza non ci capisce, e qualcuno la risposta dovrà darsela, prima o poi. Io credo che l'approvazione dell'emendamento del collega Bosone interpreti in modo preciso e puntuale il senso che abbiamo inteso dare alla *ratio* di questo provvedimento, a questo percorso. Al collega Marino e al collega Cosentino, che invitano a raccolta i medici come se fossero destinatari di un provvedimento vessatorio, io posso affermare esattamente il contrario, perché i medici attendono di esprimere il proprio convinto plauso per un testo che, già così come è, apprezzano in modo convinto e diffusissimo. e diffusissimo. Noi diamo il ricettario del Servizio sanitario nazionale a tutti i medici che operano nell'ambito di questo comparto così delicato, in modo tale che che quegli aspetti burocratici che abbiamo vissuto in modo assolutamente incomprensibile, con ripercussioni sui livelli di efficacia dell'assistenza al paziente (in particolare al paziente terminale), trovino una parola conclusiva e facciano parte ormai della storia e di una cultura che è superata. Questo è il senso, non soltanto dell'attenzione destinata agli operatori della sanità e prioritariamente ai pazienti, ma anche il senso complessivo di questo disegno di legge che merita, almeno per un minuto, un momento di pacificazione all'interno di quest'Aula, dove credo dibattito serva a formare in modo più solido il convincimento rispetto al merito e al contenuto delle leggi, piuttosto che a divagazioni di altro tipo che molto spesso portano portano fuori dalla logica che ci mette in collegamento con la nostra comunità nazionale. *(Applausi Signor Presidente, non ho compreso bene, ma ricordo perfettamente - d'altra parte mi veniva adesso sollecitato

questo sia un emendamento nodale rispetto al significato stesso del disegno di legge, la semplificazione delle terapie. Mi stupisce il parere della Commissione bilancio in questo caso l'aumento delle spese è relativo, al limite, alla carta con cui si stampano i ricettari, perché in realtà non andiamo sicuramente ad ampliare la platea dei pazienti. Sono pazienti in condizioni estremamente gravi, Stiamo parlando di pazienti terminali e di prescrizione di morfina e non di farmaci accessori, vitamine. Siamo parlando di prescrizione di morfina, di farmaci antidolore in pazienti terminali. Il significato di questo emendamento era quello di potenziare la legge in termini di semplificazione, cioè di dare il ricettario a tutti i medici che si occupano di questo materia in questo settore. Penso che questo sia davvero tant'è vero che c'era un parere favorevole da parte di tutto il Senato, opposizione, maggioranza e Governo. Pertanto, non mi sento francamente di ritirare questo emendamento. Non penso che ci sia un problema vero di copertura finanziaria né penso che il Capo dello Stato si fermi di fronte a questo emendamento, che semplicemente amplia di poco la platea dei medici, e non dei pazienti, che fanno prescrizione, semplificando la vita

identici. L'emendamento 10.202 prevede la possibilità di fare le prescrizioni dei farmaci antidolorifici nel settore delle cure palliative e della terapia antalgica.

Signor Presidente, sono costretto a replicare perché si tratta di materie di particolare sensibilità umana e sociale. Voglio rassicurare il senatore Bosone e gli altri colleghi che questi temi sono da noi vissuti esattamente come loro.

dal senatore Bosone. Ricordo che la mancanza di copertura comporta l'assunzione di responsabilità da parte del Senato di votare una norma che formalmente, secondo la Commissione bilancio, non ha copertura finanziaria, per cui poi andrà al vaglio di chi di dovere, salvo poi essere emendata dalla Camera Signor Presidente, riteniamo che l'ordine del giorno sia la formula più adatta, sia per le motivazioni addotte dal presidente Azzollini, che porterebbero al rischio di vedere annullato tutto lo sforzo fatto dalla Commissione e da quest'Aula, ma anche per un motivo aggiuntivo di carattere tecnico. In realtà, questo emendamento è pleonastico pleonastico in quanto già la legge al suo interno prevede la possibilità da parte dei medici di base e di tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale

impone una tracciabilità severissima della ricetta, ma permette a tutti i medici di prescrivere farmaci antidolorifici ai propri pazienti. Ricordo che in questo momento il 95 per cento dei pazienti oncologici in Italia non riceve adeguata terapia per il dolore e il 42 per cento dichiara che il dolore che affrontano è intollerabile. Io credo che ogni medico

grazie all'azione di tanti legislatori, il medico invece è a carico del Servizio sanitario nazionale e, come lei sa, prodotti quali il Temgesic ed altri sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Confermo, pertanto, il mio parere contrario

e, nei fatti, producendo una legge difficilmente comprensibile a una prima lettura. Questo, però, è ciò che abbiamo fatto fino ad oggi e, quindi, mi sono inserita anche io. Cosa è questo articolo 83?

gli illeciti della produzione e del traffico degli stupefacenti, «si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico».

senso; ha solo un significato di tipo culturale, cioè incute timore ai medici per la prescrizione di farmaci stupefacenti. Nei fatti, il timore di poter essere incriminati per eventuali contestazioni di un uso non terapeutico del farmaco può limitarli nello svolgimento della loro attività e quindi riduce la possibilità di

22". È stato respinto l'emendamento che prevede la prescrivibilità di questi farmaci sulla ricetta bianca, e dunque non a carico del Servizio sanitario nazionale, con la motivazione nobilissima - che ci ha dato il collega De Lillo

che né con la ricetta bianca né con quella rossa potremo dare i farmaci che servono. È francamente una specie di risultato paradossale *(Applausi dal Gruppo* *PD)*, anche per le intenzioni perfettamente condivise dalla maggioranza, che voleva una legge che consentisse, con tutti i controlli necessari, di andare incontro al bisogno dei malati.

considerata l'assoluta condivisione relativa a questo emendamento, che fa

che possa essere valutata la possibilità almeno di una sua trasformazione in un ordine del giorno che impegni il Governo a valutare, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni, una

Presidente, l'ordine del giorno non è assolutamente vincolante: impegna il Governo a valutare la possibilità o l'opportunità

quanto costa effettivamente questa legge che l'Aula del Senato afferma essere una delle più importanti di quelle approvate negli ultimi tempi? Questa legge costa 50 milioni di euro, perché la copertura che viene data, di almeno 100 milioni di euro, va in realtà a sostituire il decreto-legge n.

di cui 50 milioni almeno dovevano essere già destinati alle cure palliative, cosa che in realtà non è avvenuta per decorrenza dei termini. Quindi, a decorrere dal 2010, la copertura di 100 milioni di euro in realtà non va ad integrare,

unirmi alla sensibilità di tutta l'Assemblea nel dare un segnale in un certo senso più concreto e sostanzioso dal punto di vista della necessità di una più adeguata copertura di risorse. Un'altra considerazione, Presidente, mi consenta di

a comprendere la necessità di aumentare le risorse destinate a questo settore. Signor Presidente, stiamo parlando del potenziamento di un servizio

chiedo di poter trasformare l'emendamento 5.201 in un ordine del giorno che impegni il Governo ad uniformare, almeno dal punto di vista gestionale, le reti di terapia del dolore e delle cure palliative, in maniera tale che il servizio reso al cittadino possa essere univoco e si eviti il rischio che il cittadino debba rivolgersi un giorno ad una struttura per poter ottenere la terapia del dolore e un altro giorno

Grazie